La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 ottobre. Nella giornata di oggi non si terranno lavori di Assemblea e Commissioni in segno di lutto per la scomparsa del presidente emerito Napolitano. L’Assemblea si riunirà domani, alle ore 17,30, per la discussione generale del decreto-legge in materia di investimenti strategici. L’esame del provvedimento proseguirà nella giornata di giovedì 28 settembre. Entrambe le sedute non prevedono orario di chiusura. Il question time, previsto per la giornata di giovedì 28, non avrà luogo. Martedì 3 ottobre, alle ore 15, sarà commemorata la figura del presidente emerito Napolitano. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Il calendario della prossima settimana prevede poi la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge su iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, nonché l’esame del decreto-legge processi, incendi boschivi, salute e cultura, attualmente in discussione alla Camera dei deputati.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

mercoledì 27 settembre, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno: Discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854) La seduta è tolta